Le interrogazioni all'ordine del giorno di oggi concernono due argomenti: i vaccini contro l'influenza A e i disturbi dell'alimentazione. Su entrambi gli argomenti interverrà il ministro della salute, professor Fazio.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, quanta polemica su questa storia dei vaccini, quanta confusione sugli organi di stampa, quanta attenzione da parte delle Regioni per le loro competenze! Noi dobbiamo riflettere con attenzione su ciò che è avvenuto non solo in Italia (e su questo mi soffermerò),

c'è stata una divisione netta fra le varie organizzazioni dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, quanti erano favorevoli alla vaccinazione e quanti erano contrari. Si è sviluppato un confronto anche serrato

di dosi? La Corte dei conti ha poi sollevato critiche in merito a questo contratto che è stato assunto sulla base di un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri con i poteri di protezione civile relativi agli atti di terrorismo.

Per quanto riguarda l'influenza H1N1, dal mese di aprile del 2009 questo virus, che in precedenza si pensava appartenesse solo al genere animale, ha contagiato anche gli esseri umani; inoltre, è stata dimostrata la diffusione da essere umano a essere umano. Mi risulta che non siano ancora disponibili i dati certi per indicare quanto sia semplice questo passaggio, questa contaminazione per questo, a rischio stagionale ormai terminato, vorremmo sapere quale sia stata la sua reale incidenza in termini di decessi, focalizzando l'attenzione sull'eventuale discostamento nei confronti della normale mortalità dovuta alla comune influenza stagionale. Vorrei anche sottolineare che, dopo l'iniziale *boom* mediatico, non si è più parlato di questo virus. Mi risulta quindi scontato chiedere se, dopo l'iniziale epidemia autunnale, vi sia stata o meno la temuta seconda ondata di gennaio e febbraio. In funzione di questi dati sull'incidenza epidemica, chiedo di sapere quanti sono stati i soggetti realmente vaccinati e in quale fascia di età. Come abbiamo già sentito prima, in considerazione del precauzionale acquisto di 24 milioni di dosi di vaccino, vorremmo sapere quante sono state le dosi realmente quante sono state le dosi realmente pagate e se è andata a buon fine l'ipotesi, che era stata fatta, di vendere le dosi in eccesso ad altri Paesi. Chiedo inoltre, per concludere, se per il prossimo anno, sulla scorta dell'esperienza maturata quest'anno, non sia plausibile pensare

*(IdV)*. Signor Presidente, signor Ministro, non ripeterò ciò che hanno detto e hanno chiesto gli altri colleghi. Mi limito semplicemente a rappresentare questa "viruspatia", che ha prodotto un danno economico non solo alle casse dello Stato italiano ma, come dice il senatore Gramazio, ma anche a quelle di tutto il mondo. Questa "viruspatia", questa influenza mediatica creata ad arte (vorrei quasi dire ha consentito alle industrie farmaceutiche di raddoppiare gli utili. Oltre alla vendita di 600 milioni di dosi di vaccino, è stato calcolato che in borsa i Big Pharma in sei mesi abbiano incassato 60 miliardi di euro. Signor Ministro, vorrei anche ricordare chi c'è dietro, chi sono quelli che hanno manovrato. E allora andiamo a leggere alcune alcune cifre e alcuni dati. Chi è Vanguard? È una multinazionale. Dietro ci sono Novartis, Glaxo e Baxter; è l'avanguardia mondiale. Chi sono gli azionisti di Vanguard Group? Sono colossi come Exxon Mobil Corporation, Microsoft, General Electric, J.P. Morgan Chase, Procter & Gamble e l'immancabile Goldman Sachs.

patti leonini. E chi paga è Pantalone. Signor Ministro, io la prego di rispondere a queste domande: il costo esatto, quanti sono stati i vaccinati e quali sono i danni

che sempre più spesso il *question* *time* viene utilizzato come propaganda del Governo e non come strumento di democrazia parlamentare. Dico questo perché più volte nella Conferenza dei Capigruppo abbiamo sollecitato argomenti su cui, alla fine, si è reso impossibile il confronto. In tal senso, avremmo preferito che venisse affrontato oggi in quest'Aula il tema della pillola abortiva RU486, viste le contrapposte recenti prese di posizione dei Presidenti regionali e, in particolare, le esternazioni del neopresidente Cota. Su una cosa siamo d'accordo: noi siamo dalla parte della vita, ma è inaccettabile che vi siano differenze tra una Regione e l'altra. Su questo vorremmo sentire cosa il Governo ha intenzione di fare, e su questo mi piacerebbe ricevere una sua risposta oggi, signor Ministro. Per venire al tema all'ordine del giorno, non c'è dubbio che dobbiamo constatare che la temuta pandemia influenzale quest'anno non si è manifestata. Stando agli ultimi dati, il numero dei decessi nel mondo a causa dell'influenza suina ammonta a 17.000, cifra

I provvedimenti adottati sono stati di reale utilità nella riduzione del numero dei contagiati? Ci lamentiamo sempre tanto degli sprechi nella sanità: come accaduto anche in America,

innanzitutto che la produzione dei vaccini pandemici non differisce dalla produzione dei vaccini stagionali, in quanto ogni anno anche per gli stagionali c'è la sostituzione di uno o più ceppi.

abbiamo ordinato 24 milioni di dosi; questo anche perché l'Italia è stato il primo Paese del mondo a prendere atto delle indicazioni che all'epoca erano incerte: ci siamo presi un rischio, stabilendo che era necessaria una sola dose e non due. Noi Noi abbiamo ordinato 24 milioni di dosi, il Canada 51, la Francia 94, la Germania 50, il Giappone 54, gli Stati Uniti 251, il Regno Unito

urgenza è stata recepita dal Governo ed è stata fatta un'intenzione di acquisto di vaccino. Successivamente, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, è stato dato mandato al Ministero della salute di acquisire con urgenza il vaccino. Ricordo che nel 2005 - e qui mi riferisco a quanto è stato chiesto rispetto agli ordini preventivi, perché siamo in situazione di ordini preventivi, di opzioni - il Ministero della salute del precedente Governo aveva stipulato con le aziende Chiron,

Sulla base dei poteri delle due ordinanze (da un lato possibilità dell'esercizio dei diritti di prelazione acquisiti, che erano quelli a cui ho accennato, dall'altro possibilità di acquistare a trattativa privata), il Ministero

siamo resi conto - ripeto: è stato un rischio - che era sufficiente una dose singola. Quindi, sono state acquistate 24 milioni di dosi, per 184 milioni di euro. La Corte dei conti ha preso atto che la stipula del contratto era ineludibile e necessitata, sia per quanto riguarda le modalità e le condizioni, sia per quanto riguarda la scelta del contraente. La Corte dei conti ha altresì preso atto che i vaccini pandemici non possono essere prodotti con anticipo rispetto al verificarsi dell'evento infettivo (ed è quanto vi stavo dicendo prima) che, alla data della stipula del contratto con Novartis, non essendovi la disponibilità di un vaccino influenzale, l'amministrazione si è rivolta ad un'industria farmaceutica non solo di accertate credenziali, ma con cui era in corso una opzione di forniture. si è ritenuto opportuno inserire nel contratto la clausola che riconosce la possibilità che il prodotto venga consegnato al Ministero prima del rilascio della immissione in commercio, in quanto ciò rispondeva alla necessità per l'Italia di approvvigionarsi il più tempestivamente possibile dell'arma efficace per far far fronte al virus. Diciamo come sono andate le cose: l'epidemia è stata più leggera del previsto. Il terremoto è stato più leggero del previsto e naturalmente ci si lamenta che è stato leggero e che sono cadute poche case nonostante noi le abbiamo costruite secondo criteri antisismici. Credo che questa sia stata una fortuna per tutto il mondo. Questo, onorevoli senatori, ha causato una serie di immunità, di forme fruste

I morti quest'anno sono stati circa 250, e quindi in riduzione rispetto a quanto avviene per le normali pandemie influenzali. Ciò verosimilmente perché questo tipo di pandemia ha "seccato" (sono fenomeni epidemiologici che avvengono in immunologia) i normali virus influenzali. È stato vaccinato un milione di persone e per i prossimi anni i contratti modulari saranno fatti come in passato. La cosa

milioni di dosi sono ancora nelle Regioni in vari tipi di confezionamento, e in questa fase si sta facendo una ricognizione per recuperarle. Due milioni e mezzo di dosi sono state date all'OMS a vantaggio dei Paesi in via di sviluppo,

intende ottenere un indennizzo per il pregiudizio sofferto in relazione ai precedenti impegni contrattuali e quindi sono in corso delle trattative per addivenire in tempi brevi ad adeguate soluzioni anche riguardo a quest'ultimo aspetto.

chiarito i modi e i termini con cui si è mosso il Governo davanti a questa epidemia. Mi è piaciuta la battuta del Ministro

nei limiti che conosciamo. Dunque, ancora una volta, come ho segnalato all'inizio, il Governo italiano si è ben comportato e, a differenza di altri Governi, è riuscito a risparmiare di più perché ha speso di meno,

sanitari), mi ritengo pienamente soddisfatto dell'intervento del Governo oltre che delle risposte che il ministro Fazio ci ha dato.

quale la difficoltà era sicuramente quella di dosare il grado di protezione e quindi di individuare il numero di dosi di vaccino da acquistare. Si è fatta la scelta di comprare 24 milioni

signor Ministro, il Gruppo dell'Italia dei Valori è insoddisfatto delle risposte che ci sono state date. Dietro le legislazioni d'urgenza si nascondono i più gravi misfatti - lo abbiamo visto - e mi spiace che sia stato il doloroso terremoto dell'Aquila. Lei, signor Ministro, non ha risposto su un contratto capestro che danneggia la fiscalità generale, quindi i cittadini, né ha risposto su un conflitto di interesse latente. Almeno l'OMS sta valutando la posizione dei suoi *advisors* scientifici, molti dei quali sono consulenti strapagati delle case farmaceutiche: a Londra 11 dei 20 membri (professori universitari) che gestiscono l'emergenza sanitaria sono sotto inchiesta. Non ha neppure risposto alla domanda sugli azionisti di Vanguard ed in merito a quella Goldman Sachs che tiene le redini dell'economia mondiale e strapaga anche i Governi come consulenti.

del disastro della campagna vaccinale contro il virus H1N1 e, naturalmente, l'Italia non si è sottratta a questa colossale speculazione. Ma mi lasci dire la mia delusione nel constatare che nessuna risposta è stata data per quanto riguarda l'altro tema, quello della RU486. Vorrei sensibilizzare a questo riguardo la Presidenza affinché lo strumento del *question time* torni ad essere una delle modalità attraverso cui il Parlamento esercita la sua alta funzione di controllo su materie specificamente individuate dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e non sia una cassa di risonanza per un'opera di divulgazione dell'Esecutivo su questioni che vengono prescelte dallo stesso Governo. **Saluto

L'attenzione che l'Istituto superiore di sanità rivolge in questo campo è sicuramente importante: è infatti sotto gli occhi

Questo piano deve essere non solo di ricerca, ma anche di cura - ormai si presenta il problema dei grandi obesi - e di reinserimento di queste persone, che molto spesso vengono emarginate dalla società e dal lavoro e hanno difficoltà di movimento e persino di cura, modo di sentire nel corso della discussione che abbiamo aperto nella Commissione igiene e sanità del Senato. Dunque, vorrei chiedere, molto brevemente, che fine ha fatto il programma europeo "Guadagnare salute", che è stato avviato con il Governo Prodi nel 2007 e che aveva come obbiettivo quello di rendere facile e accessibile una serie di informazioni riguardanti proprio la correttezza nell'alimentazione, e quali sono i primi risultati del programma di monitoraggio «OKkio alla SALUTE», che è stato avviato dall'Istituto superiore di sanità

nei confronti di tali patologie le strutture sono ancora veramente pochissime, assolutamente insufficienti e poco specializzate per contrastare patologie sempre più incidenti nella nostra società.

Signor Presidente, signor Ministro, con questa interrogazione noi senatori dell'Italia dei Valori vogliamo concentrare l'attenzione sua e dei colleghi su due temi a nostro giudizio assai importanti, perché costituiscono un veicolo spesso tragicamente efficace per la diffusione di vere malattie sociali, quali sono ormai l'anoressia e la bulimia. Innanzitutto, chiediamo di sapere cosa il Governo intende fare al fine di assicurare una seria regolamentazione e un attento controllo sulla cosiddetta industria della dieta, quel vasto mercato per la realizzazione di prodotti e programmi dimagranti, ormai reclamizzati con sempre maggior diffusione, che promettono - non raramente a sproposito perdite di peso rapide e senza sforzo. L'assunzione di tali prodotti - che, nel migliore dei casi, può risultare inutile, se non accompagnata da abitudini alimentari corrette e da attività fisica - può diventare addirittura assai nociva, se posta in essere da soggetti già sottopeso, anziché con un effettivo eccesso ponderale. In secondo luogo, chiediamo di sapere se non si ritenga necessario porre in essere una regolamentazione dei siti cosiddetti pro-ana, che fanno propaganda al disturbo anoressico e bulimico e il cui numero solo in Italia si aggirerebbe intorno a 300. Voglio essere molto chiaro: noi dell'Italia dei Valori su questo punto siamo contrari a qualunque strumento giuridico che tenda a limitare la libertà della Rete, che consideriamo uno spazio prezioso; allo spesso allo spesso tempo, tuttavia, riteniamo che l'istigazione via *web* a pratiche di fatto autodistruttive, come l'anoressia e la bulimia, vada nettamente contrastata. Chiediamo dunque di sapere cosa il Governo intenda fare

alimentare sono in continua crescita, interessando circa il 15 per cento degli adolescenti. In Italia, a tutt'oggi, esistono pochissimi centri specializzati all'interno degli ospedali o di altre strutture pubbliche, la conseguenza che gran parte di questi pazienti è costretta a rivolgersi a centri privati, i quali però a fronte della spesa non sempre offrono la garanzia di trattamenti qualificati. Considerando la diffusione del problema, il Governo è disposto a rispondere a questa crescente necessità con la creazione di nuovi centri specializzati diffusi su tutto il territorio nazionale? Inoltre, parlando di obesità infantile, altro fenomeno in grande aumento, è disposto a prendere

per quanto gli interroganti hanno chiesto, cioè il discorso di portare questi aspetti nelle scuole e quindi di verificare gli aspetti educazionali. Vorrei ricordare che l'obesità ha un doppio fattore genetico, un fattore per così dire genotipico, cioè insito

«OKkio alla SALUTE» ha dimostrato è la sedentarietà dei giovani: molti giovani non fanno regolare attività sportiva; un giovane su quattro ha una televisione in camera.

Il problema dei disturbi del comportamento alimentare interessa il Governo, interessa il Ministero della salute, interessa il Ministro della salute, interessa me personalmente. È un problema importantissimo perché, al contrario di quanto molti pensano, non è un problema di cibo: è una malattia mentale. Di fatto è un problema psichiatrico, è un problema di compulsività. Da questo punto di vista abbiamo attivato (è un fatto recente, per cui non ci sono ancora delle notizie stampa) un tavolo con il ministro Meloni proprio riguardo al contrasto della diffusione di anoressia, bulimia ed altri disturbi del comportamento alimentare dei giovani. Questo filone di pratiche di cura è stato finanziato dal Ministero della salute con 300.000 euro e dal Ministro per la gioventù con 100.000 euro, mentre altri 500.000 euro sono stati finanziati dal Ministro della gioventù per la prevenzione sociale di questo specifico problema della bulimia e dell'anoressia, quindi del comportamento alimentare. Vorrei darvi anche qualche risultato di questo discorso, perché gli obiettivi erano la ricognizione dell'esistenza in termini di rete assistenziale (mi riferisco a quanto chiedeva la senatrice Bianchi), la sorveglianza epidemiologica del fenomeno, la formulazione di un protocollo di buone pratiche cliniche

in queste strutture una cosa è offrire dei servizi di consultorio, dei servizi psichiatrici, di supporto, altra cosa è semplicemente avere una residenzialità. Sono aspetti diversi, che vanno retribuiti in modo diverso e che vanno evidentemente affrontati in modo diverso. La mappa delle strutture assistenziali è stata completata e condivisa con le Regioni; questo è un primo importante risultato che il Governo ha ottenuto. Questo verrà divulgato attraverso i siti del nostro Ministero e del Ministro per la gioventù e sarà oggetto di specifica comunicazione alla stampa, ma vorrei comunque anticipare, visto che la sede

centralmente presso la Regione coordinatrice, che è l'Umbria. È partito il *follow-up*, e oggi ci sono le prime elaborazioni delle informazioni sulla tipologia dei trattamenti. È anche in fase di avanzata realizzazione il documento sulle buone pratiche di cura che va proprio ad interessare un problema di una rete nazionale. È allo addirittura pensando - ed è possibile, adesso dobbiamo verificare con il Dipartimento della programmazione sanitaria - alla eventualità di inserire un'attività specifica sui disturbi del comportamento alimentare negli obiettivi del Piano 2010, e quindi di finanziarla specificatamente per le Regioni. Ciò, per dire l'interesse che questo problema rappresenta per il nostro Governo. Il filone della prevenzione, finanziato

alle buone pratiche di cura e prevenzione sociale dei disturbi del comportamento alimentare. Sono in esso contenute tutte le delibere delle singole Regioni che sono già intervenute in questo campo.

si concluderà la discussione dei disegni di legge riguardanti l'obesità grave, in cui si parla anche di prevenzione, ci sia finalmente la relazione tecnica del Governo e che questa sostenga detta iniziativa.

attiene al diritto alla salute ma anche, in termini di strategia futura, al contenimento della spesa pubblica: più persone sane significano meno spese per la sanità. Ringrazio anche il Ministro della salute, professor Fazio, per la disponibilità e dichiaro così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno. Onorevoli colleghi, è trascorso un anno dal terribile terremoto che, nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 aprile 2009, ha investito la città dell'Aquila e la sua provincia. Tutta l'Italia, in quelle tragiche ore, si è commossa di fronte al numero impressionante di vite spezzate dalla violenza del sisma. Accanto a coloro che (istituzioni pubbliche, associazioni di volontariato e privati cittadini) si sono generosamente impegnati in prima persona nel soccorso e nella ricostruzione, altissimo è stato il numero di quelli che, dall'Italia e dall'estero, hanno dato vita ad una straordinaria gara di solidarietà per sostenere gli sforzi dei soccorritori e lenire, per quanto possibile, il dolore delle vittime. Il popolo abruzzese, colpito al cuore, ha destato l'ammirazione del mondo per la forza con la quale ha saputo reagire alla devastazione del tessuto sociale, culturale e produttivo di tanta parte del suo territorio. Molto è stato fatto, in questi mesi, per restituire una casa a migliaia di famiglie, per rilanciare le attività economiche, per limitare e recuperare gli ingenti danni al patrimonio culturale di quella Regione. Occorre però continuare l'impegno per ripristinare pienamente quel tessuto sociale e culturale - dai tesori d'arte dei centri storici alle antiche chiese, dai teatri cittadini alle università che costituisce il vanto del nostro modello di civiltà e di cui nella città dell'Aquila e nei piccoli centri della sua provincia si ritrovano alcuni fra i più fulgidi esempi. Sono certo che le istituzioni nazionali - con il sostegno delle forze politiche -sapranno continuare ad accompagnare con le iniziative più opportune ed efficaci, come è stato fatto in quest'anno, il faticoso cammino dei cittadini abruzzesi verso la riconquista della normalità. Il Presidente del Senato ha inviato ieri un messaggio al prefetto dell'Aquila per rinnovare la vicinanza e l'immutata solidarietà della nostra Assemblea alle popolazioni colpite e ringraziare tutti coloro che con abnegazione, generosità e impegno hanno offerto la propria opera per la ricostruzione. Certo di interpretare i sentimenti di tutti i colleghi, rivolgo un commosso pensiero alle 308 vittime di quella immane tragedia e, nella loro memoria, vi invito ad osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento.

Signor Presidente, è passato un anno dal sisma che colpì 57 comuni abruzzesi, causando 308 vittime e lasciando senza casa 67.000 persone. Questi sono i giorni del ricordo di una notte tragica che resterà impressa per sempre nella memoria come una crepa ineludibile per tutti noi italiani. L'Italia intera si è stretta intorno all'Abruzzo: ha portato ogni genere di aiuto cercando di raccogliere le macerie, comprese quelle più pesanti, quelle che il terremoto ha lasciato nella vita delle persone. Il *post*-terremoto è stato caratterizzato da una mobilitazione massiccia, tanto più imponente quanto più spontanea e istintiva: 70.000 persone intervenute a vario titolo nelle attività di sostegno alle popolazioni colpite; circa 12.000 volontari impegnati solo all'Aquila. Si è trattato di un aiuto concreto e un calore che è continuato nei mesi successivi e che, grazie a Dio, ancora s'avverte. Sì, perché la crepa maggior il sisma l'ha aperta nella vita della gente; ed è proprio la vita di chi è sopravvissuto ma che, tra le mura delle case crollate, ha lasciato un fratello, un genitore, un figlio, che ha bisogno di essere sostenuta concretamente e, insieme, di essere motivata. Abbiamo il dovere di non dimenticare che quelle perdite umane hanno anche compromesso il futuro di chi ce l'ha fatta, ma che non sa come andare avanti. Ciò che rende ancora più doloroso il ricordo delle vittime è dover constatare come la città dell'Aquila fatichi a tornare in vita. La sua è una rinascita fragile che dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, come non siano solo le case a fare una città. Non è ricostruendo che si ricostruisce il tessuto sociale, che si riattiva una comunità. Oggi c'è un grande rammarico guardando alla lenta ripresa delle attività lavorative: si ha in alcuni casi la sensazione di immobilità, di un clima surreale che non ha mai abbandonato L'Aquila. Abbiamo il dovere di continuare ad assicurare un futuro ad un popolo, quello abruzzese, che nel buio si è sollevato con la dignità e la caparbietà che lo contraddistingue. Tale forza deve essere ripagata innanzitutto facendo luce sulle ombre che si sono insinuate nel momento della ricostruzione: troppo spesso i quotidiani hanno riportato in prima pagina notizie di appalti truccati, funzionari pubblici collusi, presunte inadempienze della protezione civile. Il modo migliore per commemorare chi nella notte tra il 5 e il 6 aprile di un anno fa ha perso la vita è fare chiarezza, garantire giustizia e correttezza nei lavori che stanno permettendo a una Regione di rimettersi in piedi. Il modo migliore per ricordare quel dramma è impedire a certi personaggi di arricchirsi a spese del dolore di un popolo.

presunte e della rabbia manifestata anche da quel gruppo di persone che durante il primo anniversario del sisma si sono distaccate dalle oltre 25.000 che stavano marciando in silenzio. La loro protesta non deve restare inascoltata; le loro voci si sono unite per gridare che oltre ai danni materiali ci sono quelli morali, che bisogna necessariamente riparare. Dando di nuovo alle persone un tetto sotto cui abitare si può mettere una toppa sulla crepa aperta dal sisma, ma c'è un'altra ferita ed è quella che più sanguina: è l'idea che in giro ci siano ancora delle persone responsabili di quella tragedia e che forse in questo momento stanno costruendo da qualche altra parte avendo il il risparmio come unico criterio. È anche questo che, ad un anno dal sisma, non fa chiudere occhio agli abruzzesi, causando persino nei bambini crisi di panico, come hanno testimoniato alcuni psicologi che si sono trovati sul posto in questi giorni. Mi domando se il Governo abbia coscienza di quanto ancora ci sia da fare, non soltanto in termini materiali, perché neanche rimettendo in piedi l'ultima abitazione si potrà archiviare come caso risolto la calamità dello scorso anno. Se i giorni del ricordo sono anche quelli del bilancio si deve prendere atto che da quelle macerie e da chi ci passa accanto ogni giorno a un anno di distanza si solleva ancora un sussulto, che in alcuni casi si trasforma in un grido: è una forte richiesta di giustizia che nessuno si può permettere di non ascoltare. Gli abruzzesi hanno le loro ferite da guarire, le altre devono essere guarite dallo Stato ed è ora che si inizi anche a curare queste.

ad un anno da quel tragico evento del 6 aprile 2009 che ha provocato 308 morti, 1.600 feriti, tanti gravissimi danni, tra i 10 e i 15 miliardi di euro, dopo la manifestazione delle carriole organizzata dagli abitanti della città, addirittura schedati e denunciati perché colpevoli di chiedere la rimozione delle macerie del centro e la ricostruzione delle loro abitazioni, non bisogna solo piangere i morti. Al 22 gennaio 2010 il numero degli sfollati risultava pari a 10.128, di cui 1.123 nelle caserme di Coppito e Campomizzi, 8.905 presso strutture alberghiere; vi sono poi 12.056 persone che hanno avuto una sistemazione nelle C.A.S.E. Un anno dopo, i numeri del lavoro fatto in Abruzzo dalla Protezione civile sono imponenti: 70.000 persone intervenute a vario titolo nelle attività di sostegno alla popolazione colpita, con 5.957 tende, 107 cucine da campo, 47 posti medici avanzati e un ospedale da campo; sono stati costruiti oltre 150 edifici antisismici che danno un tetto a 15.000 persone e casette in legno per altre 2.000-3.000. Io sono abruzzese, ma a questo buon lavoro della Protezione civile si contrappongono purtroppo anche lo scandalo micidiale dell'inchiesta sui grandi appalti smascherata dalla procura di Firenze, le inchieste del settimanale «L'espresso» sulla gestione della Croce Rossa, l'allontanamento di alcuni servitori dello Stato come il maresciallo Lo Zito, l'immagine deleteria dei funzionari pubblici legati ad Angelo Balducci che fanno incetta di regali ed *escort* a spese di imprenditori compiacenti e della collettività, lo stridore delle risate tra le coperte pensando ai nuovi affari del terremoto aquilano ed ai nuovi appalti. Nei giorni scorsi il Capo dello Stato ha ringraziato la Protezione civile e anche noi dell'Italia dei Valori siamo grati alla Protezione civile per quanto è stato fatto, ai Vigili del fuoco e ai semplice volontari, rimarcando però che questo specialissimo dipartimento della Presidenza del Consiglio è chiamato a fronteggiare le calamità naturali e ad esse deve dedicarsi, senza perdersi in altre direzioni di intervento pubblico per ovviare alle lentezze di procedure ordinarie non ancora rinnovate e semplificate come è necessario da tempo. Non è la prima volta che il Presidente della Repubblica richiama lei, signor sottosegretario Guido Bertolaso, a dedicare le sue energie alle calamità, che sono il *core business* della Protezione civile, senza lasciarsi invischiare in altre emergenze, che poi, a ben vedere, emergenze non sono. Cosa c'entrano con la Protezione civile i cantieri per i mondiali di nuoto, per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia o per la costruzione di un *auditorium* a Firenze? Certo, in Italia le procedure sono quelle che sono e la scorciatoia di adoperare le ordinanze di protezione civile (il famoso «metodo Bertolaso») è stata fortissima, sia ai tempi del Governo Prodi, sia con il Governo Berlusconi. Quanto però quella scorciatoia fosse deleteria e foriera di guai lo raccontano le inchieste dei magistrati di Firenze e di Perugia. Dai primi di febbraio sono in carcere tre alti dirigenti pubblici e un imprenditore (un gruppo ribattezzato «la cricca» dal gip di Firenze), che sono chiamati a rispondere di corruzione. Chiudo, signor Presidente, citando Antonietta Centofanti, animatrice dell'associazione «Vittime della casa dello studente» (c'era anche Ivana Lannutti sotto quelle macerie; ci sono inoltre i giovani che hanno manifestato davanti a Palazzo Chigi, con civiltà e dignità, portando le foto dei propri cari, senza essere neppure ricevuti dal Palazzo: noi c'eravamo). Dice Antonietta Centofanti: «Dov'era la Protezione civile? Dov'era lo Stato? Non voglio pensare che in quei giorni si era troppo occupati a gestire il G8 della Maddalena, che poi aveva altri scopi».

6 aprile 2009 la notizia del terribile terremoto che aveva colpito L'Aquila e i paesi limitrofi, causando 308 vittime e 70.000 sfollati, scuoteva profondamente i nostri connazionali all'estero, in particolar modo la numerosissima comunità degli abruzzesi sparsi nel mondo. Ricordo che nella sola regione francofona della Vallonia, in Belgio, ci sono tre sindaci, italiani residenti all'estero, di origine abruzzese. Tanti si sono precipitati al telefono per avere notizie dei propri familiari o amici in Abruzzo, senza ricevere risposta. Molti, colti di sorpresa nei luoghi di vacanza (in cui si erano recati per le celebrazioni pasquali), sono rientrati anzitempo per organizzare raccolte di fondi tra i corregionali e non solo. Il sisma dell'Aquila ha avviato una corsa alla solidarietà senza precedenti, segnando un primato di vero spirito di fratellanza e di collaborazione a livello internazionale, nel quale gli italiani all'estero si sono distinti. Ecco perché, in occasione del primo anniversario del devastante terremoto, vorrei ricordare non soltanto l'angoscia e il dolore dei tanti abruzzesi residenti all'estero, ma anche la partecipazione commossa ed affettuosa di tutti gli italiani all'estero alla tragedia che ha colpito i loro connazionali abruzzesi. Vorrei inoltre che non venisse dimenticato l'impegno fattivo e concreto assunto dalle nostre comunità all'estero per alleviare le sofferenze e i disagi della popolazione e per contribuire alla ricostruzione. Tutte le comunità di italiani residenti all'estero e le varie associazioni

istituendo appositi conti di solidarietà finalizzati a raccogliere i fondi destinati alla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto. È stato detto che,

è stato ferito ed inevitabilmente sarà segnato da una cicatrice indelebile per gli anni a venire, ma il nostro Paese ha dimostrato in questa occasione un encomiabile senso di responsabilità e solidarietà. La macchina della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e delle Forze armate ha saputo gestire l'emergenza con risultati sorprendenti, riconosciuti da tutti a livello internazionale. Basti pensare che la prima scossa è avvenuta alle ore 3,32 di lunedì 6 aprile e che già alle ore 3,35 la sala operativa della Protezione civile era attiva. I primi soccorsi erano operativi di lì a poco e in serata erano già state montate 5.000 brande nelle tende e 15.000 persone erano state sistemate negli alberghi sulla costa. Nei primi due giorni dopo il terremoto erano attivi sul campo 12.000 soccorritori: pompieri, Forze armate, volontari, vigili urbani, addetti a elettricità, telefoni e strade. Nei giorni immediatamente successivi al sisma sono state predisposte 41 aree di ricovero e 17 presidi sanitari, con più di 1.600 operatori, tra cui 60 psicologi; sono state assistite 21.000 persone.

il Governo abbia preso per mano gli abruzzesi e li abbia aiutati a rialzarsi, anche mettendo la città dell'Aquila al centro dello scenario mondiale portando l'evento G8 proprio in quella terra martoriata. Un'infinità di persone provenienti da tutto il Paese si sono messe a disposizione volontariamente per portare il loro contributo alle comunità cittadine abruzzesi. Provincia e dei Comuni, ha fatto fronte alle necessità di assistenza delle oltre 70.000 persone sfollate, procedendo ad una attività di costruzione di nuove strutture, permettendo agli abitanti dell'Aquila e degli altri centri più piccoli di poter tornare subito in casa e di iniziare nuovamente il cammino verso una vita normale. In tempi rapidi sono stati ripristinati i servizi essenziali, primo fra tutti la scuola, facendo sì che gli studenti aquilani e dei paesi limitrofi non perdessero l'anno scolastico. Sono state inoltre adottate misure straordinarie per i lavoratori autonomi, soprattutto nel settore agricolo: è stata prevista la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e del premio delle assicurazioni contro infortuni e malattie professionali; è stata prevista la continuità dei pagamenti da parte degli enti previdenziali e assistenziali; è stata prevista un'indennità di 800 euro mensili a tutti i titolari di attività commerciali, produttive, agricole, artigianali e simili, che hanno dovuto sospendere l'attività per gli eventi sismici. È stata prevista la rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito e l'apertura di specifici conti correnti bancari sui quali versare i proventi delle donazioni e degli atti di liberalità da impiegare a favore delle popolazioni colpite; dei termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas. Terminata, però, ora la fase dell'emergenza saranno le istituzioni abruzzesi e aquilane a doversi far carico delle decisioni da adottare, della definizione delle priorità, sempre però con la supervisione del Governo, in modo tale che si possano perseguire anche nella fase della ricostruzione, che inevitabilmente durerà diversi anni, gli stessi risultati record che hanno permesso di attutire attutire il colpo inferto dal terribile terremoto del 6 aprile. In conclusione, il primo impegno del Governo deve essere quello di assicurare le risorse necessarie alla ricostruzione affinché quest'azione in favore delle popolazioni colpite dal sisma continui a tradursi in risultati concreti.

pertanto, anche perché non ci siano equivoci sul giudizio che noi diamo - e che a me è capitato di dare anche altre volte - su questa prima fase del lavoro rispetto alla tragedia che ha vissuto la nostra regione, la mia regione,

che ha confermato come l'Italia nel campo della struttura di protezione civile sia forse uno dei Paesi meglio organizzati del mondo. è un intreccio tra competenze statali e quest'area straordinaria che mette assieme 1.300.000 volontari dagli Alpini, che cito per primi per ovvie ragioni, all'area del volontariato cattolico - la Croce rossa per lo Stato, i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine addestrate. La struttura, guidata dal dottor Bertolaso, ha funzionato in quei momenti in maniera assolutamente straordinaria. La raccomandazione del Capo dello Stato ed anche le decisioni, faticose, che abbiamo preso in sede parlamentare, nel senso di dare a questa struttura compiti precisi che siano quelli di far fronte alle emergenze, vedrete che non sarà una scelta sbagliata; perché allargare le può toccare l'efficienza, la forza di una struttura che funziona. Secondo: intendo dare un riconoscimento a tutti, anche a me stesso, all'opposizione, agli enti locali, ai sindaci. Qual è stato nei primi due mesi di questa tragedia l'argomento che ci fece discutere di più, la questione che visivamente veniva sotto gli occhi? Noi toccammo un picco di 35.000 persone nelle tende: un'enormità.

Io ero pessimista, tanto è vero che in un dibattito televisivo una gentile signora, Ministro della Repubblica, diceva che aveva grande fiducia nel Governo

con soluzioni varie (le case antisismiche, le piccole case nei paesi e nei Comuni: sono 3.500 e solo una parte all'Aquila), è stato un risultato apprezzato dall'Italia e certamente degli abruzzesi e dagli aquilani.

dover dire la parola definitiva sui modi e sulla strategia della ricostruzione: c'è dunque bisogno di un sostegno tecnico straordinario. Il gruppo di missione,

Debbo dire che anche le indicazioni di massima, operative e politiche, che vengono date debbono essere più stringenti. C'è il problema dei danni collaterali, di Comuni ai margini del cratere, che altre volte sono stati considerati e che non trovano una risposta, anche in presenza di danni significativi. Qui una direttiva deve essere data: è sbagliato lasciare aperta la questione. Colleghi (voglio ricordare l'amico e collega Lusi, che siede davanti a me, e che diverse volte ha parlato di una vallata straordinaria proprio ai margini, la Valle Peligna, che qualche problema ce l'ha), se penso che è inagibile

*(PdL)*. Onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, non chiedo la par condicio con il presidente Marini, ma magari 30 secondi o un minuto in più mi potrà essere concesso, anche per introdurre una tematica che avevo, data la brevità del tempo, omesso di considerare nei miei appunti. Ad un anno dall'immane tragedia che ha colpito la città dell'Aquila, il suo circondario e l'Abruzzo intero, ci corre l'obbligo, prima morale che politico ed istituzionale,

perché il futuro degli aquilani non è un futuro di corto respiro ma traguarda certamente il prossimo decennio. E di questa impostazione sono anche grato al presidente Marini, perché ha colto esattamente il senso di questa commemorazione e di questo ricordo odierno. Le commemorazioni come questa, per la quale ringraziamo la sensibilità del presidente Schifani, sono utili e valide se tendono verso la verità ci sono però anche di insegnamento per guidare le vicende a venire. Per cui non faremmo cosa utile se in questo momento non riguardassimo lo scenario di appena un anno fa: una tragedia immane per le vittime, per le sofferenze fisiche e morali e per i danni materiali, in una città storica con un enorme patrimonio culturale e artistico, con grandi potenzialità turistiche, da conservare gelosamente e valorizzare come fondamento di memorie, valori, tradizioni, ma anche di progresso e sviluppo economico. Per non parlare della sua Università, vero motore di cultura e di ricchezza e delle istituzioni pubbliche, in una comunità investita del ruolo di capoluogo regionale,

Solo partendo da questo scenario si può comprendere come si sia parlato e si continui a parlare di un vero e proprio miracolo aquilano, certamente favorito dalla vicinanza e dalla facilità di collegamenti con la Capitale, ma anche da una risposta delle istituzioni locali abruzzesi, che caparbiamente vollero restare sul fronte del terremoto e non «salpare» verso lidi più sicuri. Signor Presidente,

In prima linea, come certamente era suo dovere istituzionale, il presidente Berlusconi con l'intero Governo, ma anche tanti rappresentanti politici ed istituzionali dell'una e dell'altra parte, a partire dal sindaco dell'Aquila e dai sindaci dei tanti Comuni colpiti dal terremoto, sia dell'aquilano che del pescarese e del teramano. Ma la risposta fu resa possibile soprattutto dall'organizzazione della Protezione civile, che tutti ci invidiano ed alla quale va tutta la nostra riconoscenza di parlamentari e di abruzzesi; un'organizzazione che mette insieme il meglio dei nostri organismi pubblici, come è stato ricordato, ma anche il meglio dell'impegno civile e sociale, rappresentato da quei tanti volontari che ci rendono, una volta tanto, orgogliosi di chiamarci italiani. Ebbene, alla Protezione civile, a chi l'ha saputa organizzare e valorizzare, a lei dottor Bertolaso - ce lo consenta - va il nostro plauso e la nostra riconoscenza; certamente, il plauso e la riconoscenza dei tantissimi che si sono sentiti amati e protetti dalla Nazione cui appartengono, che anche nei momenti più bui e drammatici non si sono sentiti abbandonati a se stessi certamente, la riconoscenza e l'affetto di tutti gli abruzzesi che hanno visto all'opera lei e gli uomini da lei guidati, in un contesto di efficiente e trasparente operosità,

sostanzialmente anche in quest' Aula e in questo Parlamento, allorché si è proceduto alla conversione del decreto-legge per L'Aquila, emanato dal Governo a meno di un mese da quella calamità, e che ha realizzato in pieno l'obiettivo del superamento dell'emergenza, anche con strumenti nuovi ed efficaci. Occorre ora guardare avanti e, prima di tutto, recuperare lo spirito di concordia che in questi ultimi mesi si è andato fortemente appannando, certamente anche a causa della vicenda elettorale ma anche, a mio parere, dell'aspettativa, coltivata da molti in perfetta buona fede, che la fine dell'emergenza coincidesse con l'inizio di un ritorno alla normalità, magari nelle stesse case abbandonate un anno fa e recuperando lo stesso ambiente ove per tanti anni si era svolta la propria vita. Così non è, così purtroppo non può essere, anche se è certo che la lunga attesa per il ritorno deve essere accompagnata da idee, progetti, strumenti, risorse, impegno e sacrifici.

ieri, o certi atteggiamenti protestatari che privilegiano la polemica per la polemica, strumentalizzando un giusto e comprensibile desiderio degli aquilani di recuperare al più presto la loro città. Ebbene, lo spirito di concordia e di coesione deve essere assolutamente ricostituito, *in primis* dalle istituzioni nazionali, regionali e locali. La scelta della nomina a commissario del presidente Chiodi e a vice commissario del sindaco Cialente va in questa direzione e fa ben sperare.

in questo caso, sarà necessario anche un intervento tecnico per far sì che quelle case distrutte o semidistrutte possano essere riportate alla normalità. Cerchiamo di mettere in campo questi interventi interventi con intelligenza e immediatezza e con la collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà. Vogliamo mettercela tutta come parlamentari nazionali

Casoli).* PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Guido Bertolaso.

di cordoglio e solidarietà, ma anche di conforto, espresse dal Presidente del Senato, nonché per i messaggi trasmessi alla cittadinanza aquilana e alla popolazione abruzzese colpita dal terremoto del 6 aprile dell'anno scorso. Non sono di origini abruzzesi,

grande collaborazione, disponibilità e unitarietà di intenti di tutte le componenti politiche, sociali ed economiche di quel territorio, ma anche di tutto il nostro Paese. Come ho ricordato ieri all'Aquila, la sfida della gestione dell'emergenza, ma soprattutto della ricostruzione della città e dei centri storici degli altri Comuni del cratere sismico, non riguarda solo gli aquilani e gli abruzzesi,

alla fine di novembre abbiamo chiuso l'ultima delle tende e abbiamo potuto disporre di tutta una serie di alloggi antisismici (con villette di legno, con affitti e requisizioni di appartamenti), che che hanno consentito di mettere assolutamente sotto controllo la situazione. Ad oggi, negli alberghi della costa risiedono ancora 1.850 aquilani, non i numeri che abbiamo ascoltato e letto in questi ultimi giorni e in queste ultime ore: tutti i dati ufficiali sono stati pubblicati anche sul sito

riguardano la gestione dell'emergenza del terremoto in Abruzzo, per quello che concerne le responsabilità statali e del Dipartimento della protezione civile.

Questo ovviamente riflette le esperienze dell'Umbria e delle Marche, del terremoto di San Giuliano di Puglia e di tutte le drammatiche tragedie che hanno interessato l'Italia in questi ultimi anni. In ossequio anche a questa condivisa linea politica, alla fine del mese di gennaio abbiamo passato le consegne al Presidente della Regione, che è diventato commissario e - come è stato ricordato - anche al sindaco dell'Aquila e al vice commissario. Con il sindaco dell'Aquila in modo particolare, avendo gestito insieme a lui le fasi della prima emergenza, avevamo deliberatamente scelto di occuparci delle persone e non del centro storico, che fu ovviamente perimetrato perché zona a rischio di incolumità per gli abitanti. Quando fummo in grado di riaprire, come promesso e come ovviamente è dovuto, l'anno scolastico, alla fine del mese di settembre, consentendo a 16.800 studenti di riprendere le proprie lezioni e dando quindi il segnale più forte, il più importante, il più decisivo nel garantire che L'Aquila sarebbe ripartita e si sarebbe liberata di questa tragedia, cominciammo ad occuparci in modo serio e concreto della vicenda soprattutto del centro storico, che è sempre stato - lo ribadisco davanti a questo autorevolissimo consesso - una competenza degli enti locali, ai quali avevamo affiancato appositamente un vice commissario nella persona dell'ingegner Sergio Basti, direttore regionale

Questa attività aveva già conosciuto un inizio di rimozione, che ci aveva consentito alla fine dell'anno scorso di liberare comunque il centro storico da 75.000 tonnellate di macerie, che comunque non erano la priorità della gestione emergenziale. Adesso questa vicenda ovviamente acquista importanza sempre maggiore, ma anche girando ieri nello stesso centro storico, oltre a ricevere nell'ambito di quel territorio una serie di manifestazioni (non nei confronti di una persona ma nei confronti di un sistema, assolutamente lusinghiere e gratificanti per quello che è stato l'impegno dei Vigili del fuoco, delle Forze armate, delle forze dell'ordine, del mondo del volontariato, della Croce rossa, di tutte le componenti) abbiamo comunque potuto prendere atto che molte attività sono di fatto già avviate. Agli enti locali non abbiamo fatto mancare neppure per un secondo la nostra collaborazione, che stiamo continuando a garantire, come faremo anche nel futuro; alla Regione, alla Provincia dell'Aquila e al Comune dell'Aquila, nel corso dei dodici mesi passati, con una serie di ordinanze, d'intesa con il Ministero del tesoro (come preferisce chiamarlo il presidente Marini), abbiamo garantito l'assunzione di oltre 300 tecnici ed esperti che, a mia conoscenza, sono ancora in servizio nell'ambito di queste tre amministrazioni, garantendo anche una prospettiva positiva per tutti i tecnici della famosa società «Abruzzo Engineering», che - com'è noto - era a rischio chiusura prima del 6 aprile dell'anno passato. Esiste quindi un pacchetto di competenze e di esperienze locali, aquilane e abruzzesi, che è nella piena disponibilità delle autorità locali. Non conosco la questione di questa struttura di missione per quello che riguarda le pianta organica, ma sono assolutamente convinto che

Signor Presidente, ho chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori, dopo aver ascoltato attentamente la relazione del sottosegretario Bertolaso, in quanto in questa commemorazione importante nessuno di coloro che è intervenuto ha giustamente mosso critiche, perché non ve n'erano, all'operato della Protezione civile nella fase dell'emergenza. Tuttavia, il sottosegretario Bertolaso, da bravo servitore dello Stato qual è, ha posto due questioni nel suo intervento, l'ultima sulla struttura di missione

Il punto vero che ha giustamente toccato il sottosegretario Bertolaso è il futuro, la struttura di missione è l'*incipit* per ricostruire. Se non è assegnato un fondo sufficiente alla struttura di missione, men che meno - signor Presidente - sono assegnati fondi per la ricostruzione, come lei ben sa e come sanno i colleghi esperti di bilancio in quest'Aula, allora ci chiediamo se stiamo commemorando soltanto la fase dell'emergenza, sulla quale *nulla quaestio*. Nessuno dice che cosa accadrà domani, Nessuno dice che cosa accadrà domani, perché fra i banchi del Governo non sono presenti né il Ministro dell'economia né il vice Ministro dell'economia né un Sottosegretario fra i tanti nominati all'economia che possano assumersi per bocca del Governo senza nulla togliere ai rappresentanti oggi qui presenti del Governo - la responsabilità dei fondi destinati alla ricostruzione delle abitazioni e dei luoghi di lavoro, dei danni diretti e indiretti - come li ha chiamati il presidente Marini - di tutte quelle località all'interno e all'esterno del cratere che hanno subìto danni. Le chiedo, signor Presidente, di dare se possibile

un impegno che obbligasse il Governo ad assumere - all'infinito - un provvedimento che destinasse certezze di fondi per il futuro della ricostruzione e non per l'emergenza. L'intervento del L'intervento del sottosegretario Bertolaso è inappuntabile da questo punto di vista, così come quello dei colleghi senatori intervenuti in questa sede. Manca però la parola del rappresentante del Governo che impegna i fondi, che è il Ministro dell'economia e che oggi non è presente. Le chiediamo, signor Presidente, di invitare il Governo a

però, solo ricordare che dall'approvazione del decreto-legge Abruzzo sentiamo risuonare il ritornello della mancanza di fondi e di finanziamenti anche per l'emergenza ‑ allora si diceva mentre pare che la realtà e la verità siano sotto gli occhi di tutti. So già quale sarà la risposta del Ministro dell'economia, per cui non ho alcuna difficoltà, se sarà disponibile, a che ci sia un ulteriore chiarimento in quest'Aula.

Onorevoli colleghi, in data 31 marzo 2010, il Presidente della Repubblica ha trasmesso la seguente lettera: Roma, 31 marzo 2010 «Onorevole Presidente, Le trasmetto il messaggio con il quale chiedo alle Camere una nuova deliberazione, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, in ordine alla legge: "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile,

nuovamente modificata dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 2010 e definitivamente approvata dal Senato della Repubblica il 3 marzo 2010. Voglia gradire, onorevole Presidente, i sensi della mia più alta considerazione. Giorgio Napolitano».

sociali*. Signor Presidente, con riferimento all'atto ispettivo della senatrice Baio e di altri senatori, inerente la istituzione della nuova sede provinciale INPS di Monza e Brianza, passo ad illustrare gli elementi informativi forniti dal competente Istituto. In primo luogo faccio presente, con riferimento allo specifico quesito in ordine ai criteri per la costituzione di nuove sedi provinciali, che l'INPS ha provveduto, in conformità alle disposizioni della legge n. con proprie determinazioni e nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ad adeguare l'ordinamento delle funzioni centrali e periferiche delle proprie sedi ed ha definito l'articolazione delle funzioni territoriali ed i relativi modelli organizzativi. Ciò al fine di ottenere un accentramento qualificato dei processi contabili e di gestione delle risorse umane, tenendo conto delle esigenze del territorio e dell'utenza, e realizzare un contenimento della spesa pubblica. Il nuovo assetto organizzativo, che prevede lo sviluppo di un sistema coerente al raggiungimento di efficienze operative e al rispetto delle vocazioni socio-economiche locali, intende anche assicurare un raccordo funzionale con tutte le altre istituzioni presenti sul territorio. Per quanto concerne, invece, l'ulteriore quesito posto dagli interroganti, sono in grado di informare che l'Istituto ha già provveduto alla istituzione di una agenzia complessa nella nuova Provincia di Monza e Brianza, al fine di garantire all'utenza continuità nell'erogazione dei servizi. Informo, inoltre, che il 24 dicembre dello scorso anno l'Amministrazione che rappresento ha comunicato l'avvio della procedura prevista per la costituzione del Comitato provinciale nel medesimo contesto territoriale, quale iniziativa propedeutica alla costituzione della nuova sede. L'INPS, pertanto, ha reso noto di aver posto in essere i successivi adempimenti necessari alla ormai prossima istituzione della nuova direzione provinciale di Monza e Brianza.

e la celerità nella risposta alle interrogazioni diano la ragione delle interrogazioni stesse. Se fosse stata data risposta in tempi più celeri

garantire una reale e sostanziale efficienza, tenuto conto che questa zona del Paese, dal punto di vista produttivo, necessita sia della sede provinciale dell'INPS sia di tutti i servizi connessi per poter assolvere a dei compiti importanti, sia sul versante dei lavoratori che su quello datoriale. **Saluto

non esprimeva alcuna volontà politica preclusiva in ordine alla costruzione dell'aeroporto di Agrigento, bensì intendeva rappresentare, in base agli elementi forniti in merito dall'ENAC, lo stato dell'istruttoria tecnica, fase propedeutica alla realizzazione del progetto presentato dalla Provincia di Agrigento. Invero, nell'appunto, premessa l'idoneità dell'area indicata e la compatibilità delle dimensioni dell'aeroporto con le tipologie delle attività individuate nello studio, si formulavano riserve in ordine alla possibilità che la futura gestione aeroportuale fosse «in grado di raggiungere 1'equilibro economico sia per le caratteristiche intrinseche del futuro scalo sia per lo sviluppo del traffico». Con la successiva nota del 18 febbraio 2010, emessa d'ordine del Ministro, si è inteso precisare che la suddetta istruttoria risulta ancora in corso e che eventuali altri progetti saranno comunque esaminati dall'ENAC e potranno essere valutati positivamente, dato che l'equilibrio economico-finanziario è garantito, secondo quanto affermato dalla Provincia di Agrigento con la nota n. 6642 in data 18 febbraio 2010, con risorse regionali. Pertanto, come fatto rilevare dall'ENAC, non resterebbe che l'inserimento dell'opera nel piano di trasporto regionale, compatibilmente con le prescrizioni ambientali.

è rimasto diversi giorni e notti, per sua scelta, in una tenda, per protestare contro risposte che non arrivavano. Quando le parlo di 40 anni non esagero, perché deve sapere che questa idea dell'aeroporto di Agrigento, nella mitica Valle dei templi - non ovviamente

il quale prospettava la necessità di costruire l'aeroporto, magari a una sola pista, nella fascia meridionale della Sicilia occidentale. Le motivazioni che lo stesso cita le voglio riportare testualmente. Proprio in quella seduta della Camera, l'onorevole Sinesio disse: «(...) vorrei far presente al Governo la necessità di costruire un aeroporto, magari a una sola pista, nella fascia meridionale della Sicilia. A questo proposito sono già state iniziate delle indagini e degli

in quella seduta diceva: «Va tenuto presente che un aeroporto collocato nella zona da me indicata sarebbe utile soprattutto per la città di Agrigento, attualmente tagliata fuori, oltre che dalle vie di comunicazione aerea, anche da quelle ferroviarie e stradali, nonostante che in quella zona stia sorgendo una zona industriale in rapida espansione». Questo lo diceva oltre 40 anni fa. Come Sottosegretario di Stato alle infrastrutture lei saprà per quanto riguarda le ferrovie, da Agrigento centrale a Palermo occorrono 2 ore e 16 minuti, da Agrigento a Messina 5 ore e 50 minuti (oggi, non allora), da Agrigento a Catania 4 ore e 14 minuti, da Trapani a Catania per percorrere 316 chilometri occorrono da 8 ore e 26 minuti a 15 ore e 18 minuti. Per quanto riguarda i porti si deve sapere che a Porto Empedocle non è possibile far passare navi che superino i 15 metri di pescaggio: quindi navi da crociera e commerciali di un certo tipo sono Agrigento oggi è l'unica Provincia della Sicilia a non avere nessun raccordo autostradale. Quello che diceva 40 anni fa l'onorevole Sinesio ancora oggi - allo stato dell'arte - la situazione in cui versa quella realtà, mentre è opportuno cercare di avere lo strumento dell'aeroporto per far sì che la Valle dei templi, patrimonio dell'umanità, possa essere visitata

prevedeva la realizzazione dell'aeroporto della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), assieme a quelli di Napoli, Firenze e Olbia-Costa smeralda: tutti gli aeroporti vengono realizzati tranne quello di Agrigento. Nel 1971 il ministro Lauricella, che lei ricorderà bene, esprime parere favorevole sulla località Piano Romano di Licata e dà questa indicazione al Ministero dei trasporti. L'ingegner Marra, direttore dell'aeroporto di Torino, incaricato dalla Provincia regionale di Agrigento, redige il progetto dell'aeroporto di Agrigento e lo consegna. Negli anni 1976-1977, si dibatte il problema. Nel 1977, il consiglio provinciale, con la delibera n. 100 (che è rimasta famosa), approva il progetto di convenzione con il Ministero dei trasporti per la costruzione dell'aeroporto, impegnandosi anche ad una compartecipazione alla spesa, sempre nella piana di Licata a Piano Romano. Da allora (la facciamo breve), cinque progetti di fattibilità sono tutti finiti in una bolla di sapone,

realizzato. L'accordo di programma quadro per il trasporto aereo sottoscritto fra Stato e Regione nel 2001 dice: «il presente accordo sarà completato a seguito degli esiti favorevoli dello studio di fattibilità

un sacco di movimento terra, e si tornò di nuovo a Piano Romano, arriva la nota - cui lei ha accennato - da parte del capo di Gabinetto consigliere Claudio Iafolla. Ciò che ha turbato tutti è stato proprio quanto c'è scritto lì. con le tipologie di attività individuate in quest'ultimo studio, non ritiene ipotizzabile una gestione in grado di raggiungere l'equilibrio economico». Lei ha citato proprio l'equilibrio economico, sottosegretario ringraziando il Presidente, che mi ha concesso qualche minuto in più). Dove si trova l'equilibrio economico nell'aeroporto di Albenga, che ha avuto nel 2008 soltanto 1841 passeggeri?

che quanto da lei detto possa essere terapeutico per il Presidente della Provincia, che in questo momento ci sta vedendo e ascoltando dall'ospedale di Agrigento (che per fortuna è rimasto aperto, grazie all'intervento del sottosegretario Bertolaso,

(i soldi della Regione, 30 milioni stanziati, privati pronti a prendere la gestione in mano) - «non sussisterebbero presupposti e condizioni tali da poter dare seguito alla richiesta della Provincia di Agrigento». Ed ecco quello quello che succede: movimenti di piazza, sindacati che fanno manifestazioni, tutta la cittadinanza e tutta la Provincia che fanno una grande manifestazione. Ma arriva la seconda nota del dottor Claudio Iafolla, che dice: che dice: «Ad integrazione di quanto rappresentato (...)» - nella prima nota - «occorre chiarire che l'appunto che le è stato inviato costituisce una nota interna e non la volontà politica di questo Ministero».

occorre forse che venga stesa un'altra novella del nostro premio Nobel agrigentino Pirandello, o forse occorre piuttosto un'indagine del commissario Montalbano, principe ed eroe di un altro scrittore agrigentino, Camilleri?

Signor Presidente, mi riferisco all'interrogazione presentata dalla senatrice Fontana, con la quale chiede informazioni circa l'eventuale ricorso da parte del Ministero alle prerogative previste dal codice dei beni culturali per sottoporre a tutela paesaggistica l'area dei fontanili e delle risorgive in località Caravaggio, ove il piano cave della Provincia di Bergamo prevede la realizzazione di un ambito estrattivo. A tal proposito, come già fatto in occasione della risposta fornita all'interrogazione parlamentare numero 5/01989, presso l'VIII Commissione (ambiente) della Camera dei deputati, voglio anzitutto rappresentare che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

In virtù di tale trasferimento, come è noto anche alla senatrice interrogante, la Regione Lombardia (con legge n. 7 del 16 giugno 2003) ha emanato il proprio piano regionale delle attività estrattive. Ciò premesso, voglio evidenziare che non rientra tra le competenze del Ministero dei beni culturali la valutazione degli eventuali impatti idrogeologici segnalati dall'interrogante, pur considerando che, laddove l'esecuzione dei lavori del piano cave in argomento dovesse determinare un'alterazione della situazione del suolo, con danni alla falda freatica che alimenta il Sacro Fonte di Caravaggio, ciò costituirebbe sicuramente un fatto molto grave, anche sotto In questo senso, intendo assicurare che gli uffici territoriali del Ministero stanno effettuando una costante attività di controllo finalizzata alla valutazione di eventuali potenziali potenziali lesioni dei valori culturali presenti in località Caravaggio e, se del caso, all'attivazione di tutti gli strumenti di tutela previsti dal codice dei beni culturali. Preciso infine che il Santuario di Caravaggio, realizzato sul progetto dell'architetto Pellegrino Tebaldi della seconda metà del XVI secolo, è sottoposto a vincoli con prescrizioni già dal 1981 in quanto, oltre ad essere uno dei monumenti più significativi della bassa bergamasca, costituisce da sempre un luogo di fede di eccezionale importanza, che richiama ogni anno migliaia di visitatori.

tuttavia, non mi ritengo soddisfatta perché, anche se c'è un segno di attenzione al valore che il Sacro Fonte del Santuario di Caravaggio ha per il territorio,

rispetto ad un'opera che rischia di avere un impatto devastante sul territorio. Peraltro, nel frattempo, visto che l'interrogazione è stata presentata ben sei mesi fa, la giunta regionale lombarda ha reinserito la cava in località Caravaggio nel piano cave della provincia di Bergamo, nonostante il nonostante il consiglio regionale si fosse espresso a maggioranza contro e nonostante il fatto che la motivazione dell'accoglimento da parte del TAR del ricorso promosso dal titolare della cava contro la deliberazione consiliare si basasse esclusivamente su un difetto di motivazione della decisione assunta dal consiglio. E così, anziché procedere allo svolgimento di un'adeguata e approfondita istruttoria al fine di produrre la necessaria motivazione, cosa fa la giunta regionale? Inizia dalla fine e reinserisce il polo estrattivo nel piano cave. In questo caso, sì, una scelta assunta con grave assenza di motivazione, scavalcando il ruolo stesso del consiglio regionale. Sono ben consapevole che la competenza sull'approvazione dei piani cave è attribuita alle Regioni, ma ho voluto interrogare il rimango convinta che vi siano ragioni che vanno ben al di là della mera competenza regionale e chiamano in causa il ruolo stesso del Ministero dell'Ambiente, che

la prima, nei documenti e nelle comunicazioni prodotte, sia a livello nazionale sia a livello comunitario, che riguardano la pianificazione territoriale, si trovano riferimenti a quattro principi ispiratori delle scelte territoriali: quello ambientale, quello economico, quello sociale e quello del processo partecipativo. Tutti disattesi nel percorso di approvazione di quest'opera di escavazione. Voglio qui sottolineare che è un territorio intero, nelle sue diverse espressioni locali - istituzionali, sociali, ambientali, economiche e religiose ad essersi unito per scongiurare la realizzazione di un progetto dall'impatto così devastante sotto vari aspetti. Ricordo che siamo in una delle zone più pregiate della pianura padana, la zona dei fontanili e delle risorgive,

I fontanili da secoli alimentano il reticolo idrico e sono tuttora elementi di importanza strategica di ambienti ormai unici in alcune parti della pianura padana, come è quella a Nord della provincia di Cremona nella zona dell'Alto cremasco e della Bassa bergamasca. Da qui discendono per la mia terra anche le motivazioni economiche, perché si rischia di produrre scompensi socio-economici sulle attività territoriali locali, con un sensibile danno al reddito agricolo della zona, mettendo così in crisi un'agricoltura fiorente e un territorio agricolo tra i più fertili e produttivi dell'intero Paese.

Vi sono, quindi, fondate motivazioni per chiedere al Governo di intervenire, anche perché credo che al territorio sia dovuta una spiegazione rispetto ad una situazione a dir poco paradossale e certo contraddittoria: infatti, nell'approvare il progetto della BreBeMi e del suo allegato «Piano cave di prestito», il CIPE ha stralciato una cava di prestito, anch'essa inserita in località Caravaggio, facendo proprie le motivazioni rese dalla speciale commissione VIA in base alle quali si evidenzia il rischio di impatti permanenti al regime idrologico (così dallo studio del Ministero dell'ambiente). Come sono conciliabili nello stesso luogo risposte così divergenti? Ecco perché ho chiesto al Ministero di attivare gli strumenti di tutela previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Ricordo infatti che, certo, la legislazione ha delegato alle Regioni la competenza in materia di tutela delle bellezze naturali, ha stabilito che lo Stato conservi un potere di inibizione o sospensione dei lavori quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali. naturali. La seconda ragione della interrogazione riguarda la richiesta di sapere se il Ministero intenda ricorrere alle prerogative richieste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio al fine di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area dei fontanili e delle risorgive in quanto area di elevato interesse pubblico, proprio per le ragioni che ho cercato di evidenziare. Anche perché, sebbene già una legge della Regione Lombardia del 2003 impegnasse la Giunta a predisporre un progetto fontanili

sono qui ancora a ribadire ed auspicare che lo stesso Ministero, ascoltando il grido di allarme e di preoccupazione che un intero territorio in modo trasversale esprime, faccia la propria parte esercitando le prerogative cui può ricorrere per conservare un patrimonio naturalistico, ambientale e socio-economico di elevata qualità.

La seduta è tolta